Comunico che in data 22 giugno 2023 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» (774). grazie.

in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul provvedimento, si è stabilito che, successivamente, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama. L'ordine del giorno della seduta di domani prevede, altresì, la consegna del testo delle comunicazioni rese alla Camera dei deputati dal Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023. La discussione sulle stesse comunicazioni avrà luogo, sempre nella seduta di domani, a partire dalle ore 15,30. Giovedì 29 giugno, alle ore 15, si terrà il *question time* con la presenza dei Ministri della giustizia e dell'università e della ricerca. La prossima settimana sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni. L'Assemblea si riunirà mercoledì 5 luglio per l'eventuale seguito di argomenti non conclusi e, alle ore 15, per lo svolgimento di un'informativa del Ministro del turismo sui fatti connessi a un servizio giornalistico televisivo e successivi articoli di stampa. I Gruppi avranno a disposizione cinque minuti. Nella settimana dall'11 al 13 luglio saranno discussi i disegni di legge, dalla sede redigente, sui seguenti argomenti: istituzione del Museo della Shoah in Roma; Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza; agricoltore custode dell'ambiente; ripristino della festività nazionale del 4 novembre. Il calendario prevede, inoltre, il disegno di legge su disposizioni sanzionatorie per il deturpamento di beni culturali e paesaggistici. I relativi emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 6 luglio.

l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di iniziativa parlamentare già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo in materia di sicurezza sociale tra l'Italia e la Moldova, sottoscritto nel giugno 2021, che persegue l'obiettivo di facilitare il flusso di informazioni e di dati tra le istituzioni di sicurezza sociale dei due Paesi - per la parte italiana: l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) - assicurando al contempo l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale. Con la sottoscrizione di questo Accordo, l'Italia e la Moldova si impegnano ad assicurare la certezza giuridica nella tutela dei diritti legati all'attività lavorativa, in condizioni di reciprocità. Inoltre, si prevede la trasferibilità dei trattamenti pensionistici a favore di tutti i cittadini che hanno prestato o prestano la propria attività lavorativa nei rispettivi territori.

ci riportano al lavoro svolto dalla Commissione, anche con una recente visita istituzionale che è stata fatta nella Repubblica di Moldova, insieme al senatore Speranzon e al vice presidente Menia.

La questione di merito è importante, perché molti cittadini e cittadine della Repubblica di Moldova assolvono delle funzioni importanti all'interno del nostro mercato del lavoro, in particolare nell'assistenza nell'assistenza familiare e più in generale nel nostro sistema produttivo e dei servizi. Occorreva quindi assicurare una copertura di carattere giuridico a queste persone, la cui presenza è significativa. Ricordo all'Aula che è talmente forte l'emigrazione dalla Repubblica di Moldova verso altri Paesi, in particolare dell'Unione europea, che in quel contesto la definiscono, con una parola molto forte, "diaspora". Mettere sotto tutela, dal punto di vista del sistema delle relazioni e del riconoscimento delle garanzie internazionali, questo tipo di situazioni è sicuramente un interesse preminente anche del nostro Paese.

della questione specifica. È necessario, infatti, un preciso segnale a quei cittadini, ai loro governanti e ai loro parlamentari: l'attenzione del mondo occidentale sarebbe bene dire del mondo libero, visto quello che sta accadendo in queste ore sul versante Est - è vera, reale e concreta e si sostanzia sia in un'attenzione e in una solidarietà di natura politica, sia nella traduzione di atti fondamentali. Per questo motivo annuncio il voto favorevole del Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe.

Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle alla ratifica dell'Accordo con la Repubblica di Moldavia. L'Accordo persegue l'obiettivo di facilitare lo scambio di dati tra le istituzioni di sicurezza sociale, per l'Italia l'INPS e l'INAIL. L'Accordo prevede inoltre l'esportabilità delle pensioni, cosa già permessa dall'Italia rispetto ai lavoratori moldavi, ma non viceversa; quindi attuiamo il principio di reciprocità. L'Accordo prevede anche la protezione dei dati personali e va a precisare meglio i termini dimora e residenza, che nei due Stati sono intesi in maniera diametralmente opposta. Questo testo è già stato approvato dalla Camera dei deputati.

mi limito a riportare brevemente la dichiarazione di voto fatta già in Commissione affari esteri. Abbiamo l'esigenza di riportare a fattor comune tutte quei Paesi europei che non fanno parte dell'Unione europea, che ci chiedono un riconoscimento, alla luce delle numerose comunità che svolgono una serie di lavori e di professioni in Italia, che qui pagano le tasse e i contributi e che hanno bisogno di vedere riconosciuta l'esportabilità delle prestazioni o comunque che ci sia uno scambio di informazioni sempre più accurato tra gli organismi competenti e le casse contributive di entrambi i Paesi. Da questo punto di vista, lo vediamo come un avanzamento e una maggiore tutela di chi lavora onestamente, paga le tasse e i contributi e deve essere di conseguenza tutelato. Quindi esprimiamo il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico.

l'Assemblea è chiamata ad esaminare il testo unificato di due disegni di legge, entrambi di iniziativa parlamentare, uno presentato dal senatore Alfieri ed altri e l'altro dai senatori Berrino e Liris, recanti la ratifica dell'Emendamento n. 1, sottoscritto dall'Italia e dal Principato di Monaco, nel maggio 2021, alla Convenzione generale di sicurezza sociale firmata da entrambi i Paesi nel 1982. L'emendamento in via di ratifica intende modificare la Convenzione vigente del 1982 allo scopo di disciplinare il telelavoro svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Viva-RenewEurope siamo favorevoli al voto che ratifica questa Convenzione importante con il Principato di Monaco, ma non possiamo non far notare,

con il quale confiniamo, nel quale molti nostri concittadini si recano ogni giorno a lavorare e che, anch'esso, non fa parte dell'Unione europea. Sto parlando della Svizzera. Come tutti i colleghi ricorderanno, poche settimane fa abbiamo approvato definitivamente il nuovo trattato bilaterale tra Italia e Svizzera che regola anche la parte fiscale dei lavoratori italiani che si recano in Svizzera per lavorare quotidianamente e in quella sede emerse la problematica che è stata risolta cioè, alla questione della normativa sul telelavoro. Signora Presidente, è piuttosto curioso che la Repubblica Italiana decida di accordare la possibilità per i lavoratori italiani che si recano nel Principato di Monaco di svolgere due terzi del loro orario di lavoro attraverso il telelavoro,

questa possibilità, oggi assicurata ai lavoratori frontalieri del Principato di Monaco, anche ai lavoratori frontalieri che si recheranno in Svizzera; diversamente andremmo a creare una situazione di disparità. Peraltro, è stato lo stesso Governo a stabilire la data del 30 giugno come fine del termine provvisorio nel quale si poteva, a seguito della situazione previgente,

per dichiarare il voto favorevole caso si applica il principio di reciprocità tra i lavoratori e, come fatto notare dal senatore Enrico Borghi - ne discutevamo qualche minuto fa - non possiamo non rimarcare la spiacevole disuguaglianza di trattamento tra alcuni lavoratori ed altri. Tra l'altro, come è già stato fatto notare, i lavoratori italiani possono rimanere sul proprio territorio per i due terzi del proprio orario lavorativo, mentre ai lavoratori

Signor Presidente, noi abbiamo voluto riproporre la ratifica per l'esecuzione di un emendamento alla Convenzione sociale tra Principato di Monaco e la Repubblica italiana per affrontare essenzialmente il tema del telelavoro. Diversamente dalla ratifica precedente, relativa a un nuovo Accordo con la Repubblica di Moldova per tutelare i tutelare i lavoratori finora scoperti, in realtà con il Principato di Monaco abbiamo da tanto tempo una Convenzione che regola i rapporti, le prestazioni sociali, le modalità di versamento dei contributi. però ritenuto necessario insistere e spingere sulla ratifica di questo emendamento, presentandola come Partito Democratico su sollecitazione delle forze sociali, dei sindacati, del territorio (in particolare i rappresentanti istituzionali della Provincia di Imperia), perché rischiavano di essere messi in discussione alcuni rapporti di lavoro; inoltre alcuni comportamenti discriminatori rispetto alla possibilità di proseguire tali rapporti. È chiaro che, alla luce di quello che è accaduto con il Covid, un'estensione del telelavoro in quella fase ha fatto capire a molte realtà, a istituzioni finanziarie e società, che potevano organizzare il lavoro in maniera diversa, utilizzando in maniera estensiva il telelavoro. Questo porterebbe a penalizzare, dal punto di vista

dovrebbero pagare in parte alla cassa monegasca e in parte all'INPS: una complicazione per i datori di lavoro - che poi metterebbero in atto una sorta di rappresaglia nei confronti di lavoratori - e per i lavoratori stessi. È un tema - lo sollevava anche il senatore Marton poco fa - che stiamo ponendo con forza e ci aspettiamo delle risposte dal Governo con la Svizzera. Noi siamo andati a tutelare dei lavoratori, anzi non ancora, perché non è stato ancora pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il nuovo Accordo fiscale Italia-Svizzera; però ci siamo posti il problema di come tutelare, dal punto di vista del telelavoro e quindi dal punto di vista fiscale e dei contributi sociali, quei lavoratori che svolgono fino al 40 per cento del proprio lavoro sul territorio italiano e che rischierebbero di essere penalizzati. Il Governo si era preso un impegno anche sulla base di ordini del giorno approvati, ma purtroppo non li sta ancora mantenendo. I ritardi nella pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'Accordo rischiano di lasciare

In questo senso - in maniera diversa, però il principio è lo stesso - con l'emendamento in esame andiamo a tutelare i lavoratori che si muovono ogni giorno essenzialmente dalla Provincia di Imperia, ma non solo, per andare a lavorare nel Principato di Monaco,

un accordo sul telelavoro, tanto che il nostro ambasciatore a Monaco Giulio Alaimo non più tardi di due settimane fa, sentito il Ministero del lavoro, ha dovuto prorogare la Convenzione in attesa che il Parlamento - in questo caso il Senato - ratificasse la stessa. Ringrazio per la velocità dei lavori la 3a Commissione e ribadisco l'importanza di questa ratifica, che è stata richiesta dalle parti sociali che rappresentano i lavoratori italiani, ma che è molto sentita e molto attesa anche nel Principato di Monaco, viste le particolari condizioni della viabilità a Monaco e viste le particolari condizioni del trasporto ferroviario che legano la Liguria e soprattutto la Provincia di Imperia alla Francia e, quindi, al Principato di Monaco. Questa ratifica mette in sicurezza tantissimi nostri lavoratori e la sua assenza, per le grandi difficoltà burocratico-amministrative che le aziende con sede nel Principato di Monaco avrebbero dovuto affrontare, avrebbe messo a rischio gli attuali occupati.

L'adozione di questo accordo risponde, com'è chiaro, all'esigenza di regolamentare specifiche forme di assistenza giudiziaria, quali ad esempio l'audizione di testimoni o imputati attraverso la videoconferenza, nonché a rendere più rapide le procedure di cooperazione bilaterale, prevedendo la possibilità di una comunicazione diretta tra autorità giudiziarie competenti. L'articolo 3, in particolare, quantifica gli oneri complessivi dello stesso (67.835 euro) a decorrere dal 2023. dal 2023. La ratifica in argomento non presenta profili di incompatibilità, né con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea, né confligge con altri obblighi di ordine internazionale del nostro Paese. Per tale motivo la proposta all'Assemblea è ovviamente di passare all'approvazione della legge di ratifica.

Il Partito Democratico voterà sì alla ratifica di questo trattato e lo farà anche per una ragione di colore politico. Il Partito Democratico, le donne e gli uomini che animano questo movimento politico, credono fermamente nei valori in esso racchiusi. Sono quelli della collaborazione, dell'agire rapido e transnazionale che consente di dotare gli inquirenti di quegli strumenti efficienti ed attuali per combattere le mafie e in generale una criminalità organizzata che non ha alcun limite nazionale nell'agire o nell'investire o ripulire denaro. Se vogliamo combattere la criminalità dobbiamo, signor Presidente, essere capaci di mantenere il loro passo evolutivo. Per questo, la ricerca di accordi bilaterali con Paesi non appartenenti all'Unione europea diviene fondamentale. Come ci ricordavano in precedenza i colleghi, l'accordo prevede specifiche forme di assistenza giuridica, inclusa l'esecuzione di congelamenti, sequestri e confische di beni, che costituiscono proventi di reati. Colpire i patrimoni della criminalità organizzata, aggredirli lì dove fa male e dove si limita la loro azione è fondamentale. Io voglio solamente ricordare che negli anni Settanta ho avuto l'onore di collaborare con chi intuì quanto importante fosse combattere la criminalità organizzata aggredendo i loro patrimoni. Purtroppo, pagò con la vita: si trattava dell'onorevole Pio La Torre, trucidato dalla mafia siciliana. Concludo, signor Presidente, affermando che, con questo accordo, facciamo un passo in avanti nella lotta alla criminalità organizzata a livello internazionale e dotiamo le forze inquirenti di potenti strumenti in campo internazionale.

è stata giustamente caratterizzata, è chiaro che non possiamo che essere convintamente favorevoli alla ratifica di questo accordo, che ovviamente ha un unico scopo: quello di rendere più efficace il contrasto alla criminalità. Quindi, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia, perché tutte le questioni che vengono affrontate e sviluppate, che vanno a integrare la Convenzione europea del 1959, fanno sì che il rapporto tra Italia ed Armenia nel contrasto alla criminalità non può che migliorare, sperando appunto di poter diventare un mattone per arginarla ancora di più.

che vuole ratificare il protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, firmato a Ginevra nel lontano 19 maggio del 1956 e ratificato, ad oggi, da 58 Paesi. L'evoluzione tecnologica, la diffusione dell'uso delle comunicazioni elettroniche nei trasporti e nel commercio internazionale hanno portato alla stipula, nel febbraio del 2008, del protocollo addizionale alla convenzione, che è quello oggi al nostro esame, che è finalizzato per l'appunto a consentire l'utilizzo della lettera di vettura in formato elettronico. Questo, in tutta evidenza, è un modo per modernizzare il traffico internazionale di merci su strada mediante il progressivo superamento dei documenti cartacei. Il protocollo addizionale, entrato in vigore nel 2011, agevola giuridicamente l'uso delle lettere di vettura elettroniche, non modificando comunque il quadro delle disposizioni sostanziali della convenzione del 1956. In conclusione, signor Presidente, si propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

il Protocollo adegua semplicemente la Convenzione esistente, applicandola alle nuove tecnologie che sono sorte. Per chi, come me, commercio elettronico e fa ampio uso di queste tecnologie è una semplificazione e ha degli aspetti giuridici importanti. Per questo motivo esprimo il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023, deliberata dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023 (*Doc.* XXVI, n. 1); valutata

sull'autorizzazione a quattro nuove missioni internazionali per l'anno 2023. La deliberazione concerne la partecipazione italiana a quattro nuovi impegni operativi, il primo dei quali in Ucraina: l'obiettivo strategico di tale missione è quello di contribuire al rafforzamento della capacità militare delle Forze armate ucraine di rigenerarsi e di condurre efficacemente operazioni a difesa dell'integrità territoriale del Paese, entro i confini riconosciuti a livello internazionale, nonché di consentire a Kiev di esercitare efficacemente la sua sovranità e di proteggere i civili. Vi è poi una seconda missione in Libia, istituita con decisione del 2013 e da ultimo prorogata fino al 30 giugno 2023, che ha l'obiettivo di sostenere gli sforzi guidati dalle Nazioni Unite per la pace e di prestare assistenza alle autorità libiche nella creazione di strutture statali di sicurezza, in particolare nei territori della gestione delle frontiere, dell'applicazione della legge e della giustizia penale, al fine di contribuire agli sforzi volti a smantellare le reti della criminalità organizzata coinvolte nel traffico di migranti, nella tratta di esseri umani e nel terrorismo, non solo nel Paese africano, ma anche nella regione del Mediterraneo centrale. Una terza partecipazione di personale militare in Niger. La missione, istituita nel dicembre del 2022, si connota come un partenariato militare condotto dall'Unione europea al fine di sostenere il Niger nella lotta contro i gruppi terroristici armati, nel rispetto del diritto in materia di diritti umani La quarta è una missione bilaterale di supporto alla Repubblica del Burkina Faso. La missione costituisce la prosecuzione di un programma di collaborazione pluriennale strutturato con il Burkina Faso, Paese situato nel cuore del Sahel, regione africana che ha assunto un'importanza crescente per la stabilità e la sicurezza dell'Italia e dell'Europa. Per lo svolgimento delle nuove missioni e dei nuovi impegni operativi internazionali da avviare nel 2023, la delibera prevede una consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegate nei teatri operativi pari a 153 unità, con una consistenza media pari a 57 unità e un fabbisogno finanziario per la durata programmata pari complessivamente a 11,7 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il documento XXIV, n. 7, si esprime favorevolmente in merito alla proroga delle partecipazioni italiane alle missioni militari e agli interventi a sostegno della cooperazione e dello sviluppo per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso. Il Governo, nella relazione analitica, presenta un quadro degli scenari geopolitici generali, rimarcando come l'attuale contesto internazionale sia caratterizzato da una congiuntura fluida e instabile, segnata in particolare da un conflitto, quello in Ucraina, che determina ripercussioni sistemiche di ampia portata sulle fondamenta stesse del sistema internazionale. In tale quadro, l'Italia ribadisce con fermezza la sua appartenenza all'Alleanza atlantica e all'Unione europea, rimarcando altresì la sua volontà di operare nel quadro di un multilateralismo fondato sulle regole e imperniato grazie. sull'identità mediterranea e sull'attenzione ai Balcani. Da queste linee politico-strategiche discende quindi la mappa della presenza italiana nelle missioni internazionali, oltre che degli interventi di cooperazione allo sviluppo e del contributo nel nostro Paese a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione degli ambiti geografici prioritari. L'Italia, in particolare, intende agire per salvaguardare l'interesse nazionale e proteggere i suoi cittadini attraverso la realizzazione di missioni bilaterali e la partecipazione a missioni di organizzazioni, come le Nazioni Unite, l'Unione europea e la NATO, a tutela della pace e della sicurezza internazionale, con l'obiettivo di promuovere valori fondamentali di democrazia e libertà in una cornice di collaborazione internazionale aperta e inclusiva. Punto di riferimento fondamentale per l'azione italiana nel contesto delle missioni internazionali è ancora una volta l'identità mediterranea, che anche per una dimensione storica e culturale rende il nostro Paese particolarmente sensibile e attento a tutto ciò che in questo bacino e nel contiguo Medio Oriente si origina, in termini di minacce, ma anche di opportunità e di possibilità di cooperazione. In tale quadro, il documento richiama innanzitutto il sostegno al processo di stabilizzazione della Libia per promuovere un dialogo intra-libico finalizzato allo svolgimento di elezioni parlamentari e presidenziali libere, trasparenti e inclusive. Nell'ambito del Mediterraneo allargato, fattori di persistenti instabilità si registrano in relazione alla questione israelo-palestinese alla crisi siriana, aggravata dalle conseguenze del terremoto del 6 febbraio scorso che ha colpito le regioni settentrionali del Paese e alla profonda crisi sociale, economica e politica del Libano, con importanti riflessi sul piano migratorio e in termini di sicurezza anche per i Paesi europei. La relazione offre quindi una ricognizione degli impegni del nostro Paese per l'Afghanistan, nel quadro delle operazioni e missioni militari e civili dell'Unione europea, nonché in ambito di Nazioni Unite e NATO. L'impegno dell'Italia prosegue anche nei Paesi dei Balcani occidentali, attesi a una delicata fase di completamento della transizione democratica e di progressiva integrazione nell'Unione, anche per il contributo che essi possono offrire al consolidamento della pace, della democrazia e della stabilità nel vecchio continente. Fra gli accadimenti di rilievo segnalati dalla relazione in tale ambito, che inducono a cauto ottimismo, vi sono le elezioni politiche presidenziali tenutesi in Bosnia-Erzegovina lo scorso ottobre e la concessione, lo scorso dicembre, al Paese balcanico dello *status* di candidato all'adesione all'Unione europea. Particolare attenzione viene inoltre riservata dalla relazione al continente africano, dove problematiche di sviluppo si intrecciano a fattori di instabilità politica e istituzionale, correlati a sfide epocali a sfide epocali come la crescita demografica, i traffici illeciti, il terrorismo, la crisi climatica e le dinamiche migratorie. apre una nuova finestra"). Ricordo che eventuali ordini del giorno al testo delle risoluzioni approvate dalla 3a Commissione permanente potranno essere presentati entro la conclusione della discussione congiunta. Dichiaro aperta la discussione congiunta.

brevi considerazioni, con questa premessa: il MoVimento 5 Stelle non è contrario alle missioni militari, anzi tutt'altro, per l'altissimo senso valoriale che tali missioni perseguono, per lo scopo della ricerca continua della pace in aree che sono ovviamente lontane dalla parola pace.

di appoggiare e sostenere delle raccomandazioni e degli impegni che non avevano alcun torto, se non quello di essere degli impegni ragionevoli. Primo impegno. Signor Presidente, lei sa che a ottobre il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di inviare i soldati in Ucraina.

Quello che però ci rende molto, ma molto preoccupati è l'articolo 1, paragrafo 5, il quale, a proposito dell'impiego dei nostri ragazzi in addestramento ai militari ucraini, letteralmente dice questo: «La missione EUMAM Ucraina opera nel territorio degli Stati membri».

dobbiamo decidere se vogliamo impiegare i nostri ragazzi in addestramento ai militari ucraini o se vogliamo che i nostri ragazzi - come si dice in gergo militare - mettano i loro *boots on the ground*, cioè vadano al fronte. fronte. Noi chiedevamo semplicemente questo: o un'assicurazione al Governo che questa risoluzione rimarrà tale e non si andrà in area di conflitto, cioè al fronte, ma si rimane nei confini dell'Unione europea e dei Paesi membri, oppure, se questa assicurazione evidentemente nessuno è in grado di darcela, quantomeno si venga in Parlamento quantomeno si venga in Parlamento e si dica chiaramente all'Italia che le nostre Forze armate sono destinate a calcare il terreno di guerra in Ucraina. *(Applausi).* Lo si dica chiaramente, per la semplice ragione che i cittadini devono essere informati, e il luogo dove l'informazione deve esplodere e deve espandersi è proprio il Parlamento. Non possiamo prescindere dal fatto che ci sia un Governo che non può avere il mandato politico per una decisione di questo genere. Sembra passato un secolo da quando dicevamo in questa stessa Aula avremmo mandato solo delle armi difensive, che noi stavamo fornendo solo tecnologie. Non è così, signor Presidente, non è più così. Noi siamo dentro una spirale di *escalation* che non ha più fine e non avrà mai fine. La verità è che noi dobbiamo sconfiggere è che noi dobbiamo sconfiggere la Russia militarmente e il peggior torto che stiamo facendo è che ci siamo dimenticando che la Federazione Russa ha 6.000 testate nucleari. Noi non batteremo mai una potenza nucleare; potremmo solo eliminare l'umanità, se continuiamo con questa ottica bellicista supina, rassegnata.

E l'impegno economico sta crescendo: spenderemo 314 milioni rispetto ai 216 che abbiamo speso nel 2022; manderemo 3.400 uomini contro i 2.200 dell'anno scorso; manderemo 620 mezzi terrestri, cioè 100 in più rispetto al 2022, e manderemo anche una trentina di aerei, cioè il doppio rispetto all'anno precedente. davanti a questo aumento dell'impegno italiano nelle missioni NATO chiedevamo semplicemente che il Governo cambiasse leggermente la postura supina che si ha all'interno della NATO. Inoltre, pur rivendicando tutto quello che all'interno della NATO viene discusso e deciso, si può chiedere all'organizzazione un contestuale impegno diplomatico perché ci possa essere una *de-escalation* e una soluzione negoziale al conflitto? Non stavamo chiedendo il mondo; stavamo chiedendo semplicemente, da da una parte, di rimanere fedeli alle alleanze e agli accordi all'interno della NATO e, dall'altra, di spendere una parola una parola perché ci possa essere davvero un concreto, reale, efficace, vero impegno per una soluzione negoziale. Invece, nonostante tutti gli esperti militari, come i colleghi della 4a Commissione possono confermare, sostengono che non ci sarà mai una soluzione militare a questa crisi, non ci sarà mai una soluzione militare a questa crisi, noi continuiamo solo in una direzione. Sulla Libia, la missione bilaterale di supporto alla Guardia costiera presenta delle forti criticità, ma noi non ce la sentiamo di lasciare quei centri all'interno dei quali stanno accadendo fatti che vengono puntualmente riportati dagli osservatori internazionali: parliamo di gravissime violazioni dei diritti umani; tuttavia sappiamo anche che se ci ritiriamo noi, qualcuno colmerà quel vuoto; sappiamo che se noi lasciamo tutto alle forze libiche, quelle sicuramente da sole non potranno fronteggiare quelle emergenze e quello sarà motivo di una *escalation* della violenza

pieno rispetto dei diritti umani e il libero accesso dell'ONU; non chiedevamo altro che, semplicemente, il ripristino della tutela dei diritti umani, ma anche in questo caso - vi sembrerà incredibile - abbiamo ricevuto il no del Governo. In Burkina Faso sta accadendo qualcosa di veramente anomalo. Stiamo sostenendo, equipaggiando ed addestrando forze governative, ma l'Alto commissariato ONU, Amnesty International e Human Rights Watch stanno dicendo che forze governative si stanno macchiando di delitti ed eccidi di personale civile. Anche in questo caso, abbiamo chiesto al Governo di impegnarsi affinché questa missione tra i suoi obiettivi abbia anche quello di garantire il rispetto dei diritti umani. Il ministro Tajani ha risposto che questo è nella filosofia della missione, quindi non capiamo perché anche in questo caso il Governo si sia rifiutato di raccogliere tale impegno. al senso di responsabilità: queste sono le criticità, ma resta fermo tutto quello che di buono i nostri ragazzi svolgono nel mondo, non c'è dubbio su questo; su tali impegni chiediamo però che il Governo rifletta e che prevalga la ragionevolezza su una logica che ci porterà solo morte e distruzione. Signor Presidente, l'impegno italiano nello scenario internazionale, attraverso le missioni militari e gli interventi di natura civile civile nei contesti di crisi, rappresenta il contributo fattivo dell'Italia alla stabilità internazionale e la risposta a fenomeni potenzialmente pericolosi per la pace e la sicurezza. Dopo anni nei quali le principali minacce erano di matrice terroristica, legate alla radicalizzazione, all'insicurezza cibernetica e ai traffici illeciti, l'invasione russa dell'Ucraina non solo ha rimesso al centro dell'Europa un conflitto tradizionale, anche rimesso al centro dell'attenzione l'impiego fisico dello strumento militare in un conflitto tra Stati. Purtroppo non è solo questo, poiché le ripercussioni in termini geopolitici sono enormi, come enormi potrebbero essere le conseguenze, per quello che abbiamo visto in questi ultimi giorni In un contesto così complesso e volatile, è assolutamente necessario che l'approccio italiano resti saldamente ancorato a una dimensione europea e all'asse dell'Alleanza atlantica, poi degli aspetti di carattere militare e di iniziativa civile per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a cominciare da quelli delle donne e delle minoranze. In quest'ottica, come Italia siamo chiamati ad accompagnare il rafforzamento del versante NATO sul fronte orientale, cosa che questo Parlamento e i Governi che si sono succeduti hanno sempre garantito, in particolar modo dall'avvio del conflitto in Ucraina. per il rispetto che dobbiamo ai tanti nostri militari tuttora impegnati, che l'Italia contribuisca sia in ambito NATO sia in ambito di Unione europea a tenere alta l'attenzione sui Balcani, a cominciare dai Paesi candidati all'ingresso nell'Unione. Come Italia abbiamo ancora di più il dovere di sottolineare all'Europa e alla NATO la delicatezza e, per certi versi, la centralità del Mediterraneo, che è un luogo nel quale si scarica una parte importante delle tensioni che maturano nel contesto euroasiatico, dalla presenza sempre più consistente di navi militari russe alle attenzioni cinesi, al ruolo che questi Paesi provano a giocare rispetto agli equilibri del Nord Africa e degli stessi Balcani. Il Mediterraneo rischia di rivelarsi il terreno sul quale si riverberano e proseguono tensioni innescate altrove, un'altra faccia della medaglia, un fronte sul quale per storia e collocazione geografica l'Italia non può che essere impegnata in un sempre maggior protagonismo, diventando da subito portavoce nei consessi internazionali e nei contesti delle alleanze consolidate. Un diverso coinvolgimento degli organismi internazionali servirebbe, ad esempio, in Libia. L'Italia in questo momento è impegnata sul territorio libico con sei missioni promosse dal Governo Gentiloni, un lavoro prezioso che le Nazioni Unite ci chiedono di continuare ad accompagnare per stabilizzare l'area, ma è del tutto evidente che serve un cambio di passo. La stabilizzazione delle fragili istituzioni libiche non può essere solo una questione italiana: serve una missione internazionale e serve soprattutto l'Europa attraverso un piano che favorisca il cessate il fuoco, che contribuisca al contrasto della proliferazione delle armi, che promuova

di sicurezza che riguardano il nostro continente e l'Italia: una terra di passaggio per l'Africa occidentale costiera, nonché una terra potenzialmente ricca, che offre buone opportunità per lo sviluppo proprio e per le imprese italiane. Tuttavia, oggi il Sahel è aggredito da un jihadismo assai forte ed influente, da una presenza in crescita delle milizie russe del gruppo Wagner, in un contesto di estrema povertà e dove la Banca mondiale stima che, entro il 2050, 13,5 milioni di persone, tra Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger e Chad, cadranno in povertà. in Sahel, nelle varie modalità in cui si realizza, è una chiara scelta di politica estera del nostro Paese, che il Partito Democratico ha sostenuto negli anni di Governo e confermato anche con l'apertura di rappresentanze diplomatiche nella regione, con la partecipazione a iniziative territoriali come il G5 Sahel e con il significativo impegno di cooperazione internazionale verso l'area, delineando così per la prima volta una presenza italiana in Africa occidentale con una modalità costruttiva e non avversativa. Accanto all'impegno militare, deve restare alto quello connesso sul piano strategico alla fondamentale azione a tutela dei diritti umani delle popolazioni, dei migranti e dei profughi, così come è auspicata l'azione di attività multilaterali di coalizione e di carattere europeo nell'ottica della massimizzazione dell'efficacia del contributo italiano alla lotta al terrorismo e all'attività delle organizzazioni criminali dedite al traffico di esseri umani. In tal senso, destano preoccupazione il taglio delle risorse per il settore della cooperazione allo sviluppo, già approntato in legge di bilancio e che si sta ripercuotendo negativamente su tutti i soggetti che partecipano alla cooperazione italiana: le ONG, le imprese e gli enti territoriali, che hanno visto notevolmente ridotto il loro ruolo di ponte nelle relazioni tra l'Italia e i Paesi del Sud del mondo. Particolarmente grave è anche la riduzione degli aumenti previsti per l'Agenzia della della cooperazione. In conclusione, signor Presidente, la postura italiana si deve qualificare lungo specifiche direttrici, ossia Unione Europea, NATO e Nazioni Unite, come soggetti indispensabili a un intervento finalizzato a mettere in campo tutti gli elementi necessari per la gestione e la risoluzione efficace di situazioni con un enorme tasso di complessità. È necessario accompagnare l'intervento militare con un piano di infrastrutture civili e per la difesa dei diritti universali, sempre non negoziabili, in cui bisogna anche riconoscere l'importante ruolo garantito dalle organizzazioni non governative e, in molti casi, anche dai nostri attori economici. Questo deve accompagnare le missioni già in essere, ma soprattutto quelle nuove, unitamente alle ormai riconosciute capacità e attitudini del contingente italiano, che sempre più spesso, nell'impostare una missione, viene considerato - dobbiamo dirlo con orgoglio - un elemento imprescindibile dalla comunità internazionale.

Signor Presidente, permettetemi intanto di ringraziare con profondo senso di gratitudine i 7.700 militari italiani impegnati nelle missioni internazionali,

creare empatia con le popolazioni locali con cui si entra in contatto. Credo che questa sia una caratteristica di cui il nostro Paese deve essere orgoglioso. La fase geopolitica che stiamo attraversando aggiunge alle complessità che la comunità occidentale e il nostro Paese dovevano affrontare già negli anni passati - penso alla diffusione del terrorismo di matrice islamica in Africa, in particolare nel Sahel,

Voglio ribadire un concetto che credo sia rappresentativo del Governo e anche di tutti gli italiani: l'impegno per la pace

ci dice che, mentre parliamo e anche mentre si consumava un'azione volta a minare la *leadership* di Putin, la Russia continua a bombardare incessantemente il territorio ucraino e non soltanto - questo forse è il dato più importante - la linea del fronte, ma anche città come Leopoli, a 50 chilometri dal confine con la Polonia, e la stessa capitale Kiev, con cinque morti. La domanda, quindi, è che cos'è la pace e come ci si arriva. Certamente, se ci fossero un'apertura, una cessazione delle ostilità da parte della Federazione Russa o l'avvio di un tavolo negoziale,

milizia privata, la Wagner, che conta 25.000 uomini - diverse migliaia dai quali oggi, tra l'altro, sono nel Sahel

Non è neanche l'inizio della fine. Ma forse è la fine dell'inizio». Questo è per dire che sicuramente, dopo quello che è accaduto, dopo l'avanzata della Wagner, che poi si è arrestata a 300 chilometri da Mosca, qualcosa è cambiato e questo qualcosa può essere colto come spunto da parte della comunità occidentale. È evidente, infatti, che le tensioni fra Shoigu, Gerasimov, Prigozhin e lo stesso Putin sono ormai palesi e non si possono più nascondere. Allo stesso tempo, però, dobbiamo chiederci quali sono le migliori condizioni per il popolo ucraino. l'integrità territoriale sia una prerogativa indispensabile per costruire un tavolo di pace, a meno che non si voglia dire: guardiamo la fotografia sul campo; quello che la Russia ha conquistato è la base per un negoziato. Non credo che questo sia nell'interesse dell'Ucraina e certo non spetta a noi occidentali imporre una qualunque condizione. Questo conflitto ha portato a guardare al quadrante Est dell'Alleanza, come diceva prima il senatore Licheri, con uno sforzo significativo dei nostri militari: da 2.200 a 3.400 in attività di deterrenza, deterrenza, una parola che forse si ripete troppo poco spesso. La deterrenza è il fattore chiave, come lo è avere assetti pregiati (penso all'attività di *air policing* dei nostri *Eurofighter* a Costanza, in Romania, penso alla nostra brigata schierata in Bulgaria). Queste sono disposizioni che servono a tutelare il fianco Est e i confini dell'Europa orientale,

volte, dove siamo presenti in Niger, con una missione importante a Niamey, e abbiamo introdotto adesso una missione in Burkina Faso; avevamo una *task force* coi francesi, la Takuba, ma poi, purtroppo, le condizioni sul campo e soprattutto un atteggiamento nei confronti della Francia di alcuni Paesi africani hanno portato questa missione a decadere. Più in generale, penso che si debba guardare all'Africa come a un triangolo: al Nord c'è la Libia, in cui il nostro Paese è impegnato sia in ambito europeo, sia in ambito bilaterale, sia in ambito Nazioni Unite;

dove siamo presenti cercando di creare condizioni di sicurezza in un Paese martoriato da *Al-*Shabaab**, il terrorismo islamico; e ad Ovest vi è il Golfo di Guinea, dove siamo impegnati con attività di pattugliamento anti pirateria. Questo è il quadrante africano. Nel fianco Est abbiamo rafforzato la nostra presenza, come dicevo prima, poi si determina, con attività di *naval diplomacy*, la politica estera del nostro Paese, che guarda anche al Sud Est, all'Indo Pacifico, che è un territorio altrettanto importante per le crescenti tensioni con la Repubblica Popolare Cinese e con i Paesi limitrofi, in particolare con Taiwan. Lì il nostro Paese, in questo momento, ha un assetto che viaggia verso le Filippine. Si tratta del nostro pattugliatore Morosini, una nave di grande innovazione tecnologica, che rappresenta il meglio delle industrie del nostro Paese. Questo, in sintesi, per dire che il nostro impegno, al netto di una media potenza regionale, quale siamo dal punto di vista finanziario, dal punto di vista personale è un impegno molto importante. le missioni nel Mediterraneo allargato, dove siamo impegnati, ad esempio, con l'operazione Irini. Cito un'altra missione importantissima, che storicamente ci ha visto protagonisti al suo comando: UNIFIL, in Libano. Dove noi operiamo si creano condizioni di stabilità, di benessere, di crescita, di tutela dei diritti e di prosperità. Per questo credo che le missioni militari internazionali siano uno straordinario strumento di politica estera e che sia nell'interesse del nostro Paese farle crescere ed arricchirle, soprattutto per consolidare la nostra postura internazionale per difendere i nostri interessi nazionali e la sicurezza, soprattutto dell'area del Mediterraneo, che oggi è minacciata non soltanto da quello che accade in Ucraina, ma da tensioni che si rappresentano nelle nostre acque e sotto

se, per l'appunto, le missioni sono così diversificate. A me è capitato, anche nel corso degli anni passati, in altre legislature,

agli sforzi, secondo me davvero straordinari, che fanno i militari italiani in quel contesto. Anche io, ovviamente, mi sento di ringraziarli per gli sforzi che fanno. Ricordo sempre le parole dei generali che guidavano quella missione e il loro rivendicare, con totale orgoglio, il fatto di non aver mai sparato un colpo di fucile, o almeno il fare di tutto per non sparare mai un colpo di fucile: figuriamoci quindi se non comprendo le cose che vengono dette e figuriamoci se non comprendo questi elementi. Ritengo però francamente del tutto assurdo

analizzarle e fare un bilancio; discutere degli elementi positivi e delle criticità. Ritengo che questo sarebbe un modo molto serio per approcciare la materia. Invece, l'obbligo di discutere complessivamente questioni molto diversificate inevitabilmente fa utilizzare quella che in politica si chiama la categoria del prevalente. Come sapete, la mia forza politica, la componente Alleanza Verdi e Sinistra, non da oggi esprime un dissenso molto forte e molto netto rispetto alle scelte che anche il nostro Paese ha fatto, in particolare sulla guerra in Ucraina. Evidentemente, quel tipo di scelta e quel tipo di impostazione che stiamo dando, dal mio punto di vista, sono un sufficiente "prevalente" per non poter esprimere un voto favorevole e, anzi, per doverne esprimere uno contrario. Come sapete, ritengo - riteniamo che sia necessario innanzitutto affrontare una questione più generale, se posso dire così, cioè un cambiamento profondo, una discontinuità nella partecipazione alle missioni internazionali.

che conosciamo, questa discussione si fa a dicembre, perché, giustamente, in quel mese si fanno un bilancio dell'anno precedente e un ragionamento per quello successivo. Il fatto che noi, invece, questo ragionamento lo facciamo a metà anno, in qualche modo già di per sé di per sé evidenzia un elemento perlomeno di perplessità, o comunque di grande discutibilità. Eppure, il contesto geopolitico internazionale con il quale ci confrontiamo è obiettivamente di grande complessità e instabilità. Ora però, anche qui, non è che questa instabilità sia frutto del destino cinico e baro, nel senso che improvvisamente ci siamo resi conto di avere a che fare con un contesto internazionale più instabile di prima. Evidentemente questo, almeno dal nostro punto di vista, ha profondamente a che fare con il venir meno di un approccio multilaterale alle relazioni internazionali, anche di una forzatura ideologica e materiale su un sistema profondamente polarizzato, che penalizza - credo anche molto - l'esercizio del dialogo. Si pensi molto banalmente a com'è cambiato nel corso degli anni il ruolo delle Nazioni Unite, Nazioni Unite, che versano in una condizione di grande difficoltà, ovviamente non da oggi, nel senso che negli ultimi decenni già evidenziavano una situazione complessa. Purtroppo, anno dopo anno, il degli organismi sovranazionali - vale per le Nazioni Unite, ma potrebbe valere anche per l'OSCE - parla di una difficoltà e rappresenta il sintomo evidente di una polarizzazione forte. Ne discuteremo anche domani, ma è evidente dal nostro punto di vista che la guerra in Ucraina rimane il principale fattore di instabilità. Siamo molto preoccupati - l'abbiamo sempre detto in quest'Aula, anche all'inizio della guerra, ormai un anno e mezzo fa

da una campagna particolarmente insopportabile nei confronti di tutti quei mondi pacifisti che esprimevano un elemento di dissenso. Eppure, dicevamo all'epoca e diciamo ancora oggi che queste critiche e questi elementi di dissenso non hanno nulla a che fare con un sostegno all'aggressione russa, che evidentemente non c'è e che anzi ci vede fortemente critici e in totale dissenso rispetto a quello che è accaduto. Il fatto di riconoscere questo elemento di aggressione, dal nostro punto di vista, non può però farci chiudere gli occhi sul fatto che gli sforzi diplomatici che sono stati

non dovrebbe farci dimenticare di tutte le altre crisi aperte (pensiamo a tutte quelle che riguardano il continente africano). Voglio semplicemente dire una cosa su questo: l'intervento

e sostenere le operazioni delle istituzioni libiche, che peraltro vengono chiamate in questo modo un po' eufemistico, perché - come sappiamo - si tratta della Guardia costiera. Voglio dire con chiarezza che non possiamo più continuare a sostenere - com'è stato fatto in questi anni - quelle operazioni, che non sono a nostro avviso di salvataggio, ma vere e proprie violazioni sistematiche delle convenzioni internazionali. Sto parlando dei respingimenti collettivi, che peraltro sono anche vietati dalle convenzioni internazionali. Gli organismi hanno decretato in modo molto chiaro che la Libia non è un porto sicuro, quindi il ruolo che la Guardia costiera assume è quello è quello di continuare a riportare queste persone all'interno dei centri di detenzione, come abbiamo sottolineato tante volte in tutti questi mesi e anni. Consideriamo un vero e proprio circolo vizioso quello che finanziamo, perché di fatto finanziamo i centri di detenzione,

posizione molto complessa e in una particolare posizione geografica, che ne ha fatto - com'è stato detto - un importante crocevia per la circolazione delle merci e delle persone e delle persone nella regione del Sahel, nonché per gli scambi e i movimenti tra l'Africa subsahariana e il Nord Africa. L'Unione europea e alcuni suoi Stati membri, come l'Italia, negli ultimi anni hanno incrementato le loro azioni in Niger, le cui autorità dal 2015 hanno avviato politiche di controllo delle frontiere sempre più restrittive, rendendo però in questo modo molto difficoltose le vie legali. È cresciuta

che questa linea politica porti effettivamente un beneficio nella lotta ai trafficanti, ma crediamo invece, all'inverso, che finisca con l'aiutarli. Anche da questo punto di vista consideriamo le tre missioni in Niger, che hanno come filo conduttore l'assistenza alle forze armate locali, prive delle garanzie sufficienti circa l'effettivo rispetto dei diritti umani. Come vedete, ho esaurito il mio tempo, potendo citare soltanto alcune di queste missioni, quelle più significative (almeno dal mio punto di vista) o quelle sulle quali si fondano alcuni elementi di criticità. Resta però la cosa che dicevo in apertura:

con condizioni e contesti politici, sociali e militari...

a svolgere una funzione burocratica o di mero recepimento di un atto amministrativo. Il voto con il quale il Senato, fra pochi minuti, esprimerà e tradurrà in legge l'atto con il quale il Governo predispone la presenza del nostro Paese nelle missioni internazionali è di chiara impronta politica. non solo per un antico, ma sempre valido sillogismo, sulla base del quale la politica della difesa è l'attuazione di una politica estera quindi risponde all'esigenza, all'idea e alla concezione che abbiamo del nostro ruolo, della nostra natura e della nostra stessa identità in un contesto di carattere internazionale e di alleanza; ma anche perché questo elemento non è astratto, ma risponde anzitutto alla chiara definizione di una strategia di sicurezza nazionale. E non ci voleva quello che è accaduto sabato e domenica fra il Don e Mosca per farci capire qual è il livello di fragilità,

del nostro ruolo internazionale, delle nostre alleanze e della presenza dell'Italia per assicurare in questa cornice quell'indispensabile azione di sicurezza

dalla sicurezza verso altri contesti significa fare un cattivo servizio alla nostra Repubblica. Tra poche settimane a Vilnius si svolgerà il vertice della NATO, quell'organizzazione che anche in quest'Aula qualcuno vede come fumo negli occhi e che invece ci ha assicurato settant'anni di pace, di stabilità e di sicurezza. In quel vertice si prenderà atto delle cose che sto sommessamente provando a raccontare e noi non possiamo guardare da un'altra parte, né possiamo immaginare che ci sia qualcuno che fa il lavoro per noi; assumerci *pro quota* la nostra responsabilità, all'altezza del ruolo, della dignità, della storia e della tradizione che la Repubblica italiana possiede. Ecco cosa sono le missioni internazionali: non un dazio da pagare o una scelta che bisogna fare perché dall'altra parte dell'oceano c'è un occhiuto alleato che pretende di mantenerci all'interno del suo sistema di potere; le missioni internazionali servono per garantire sicurezza, stabilità e pace al nostro Paese e al teatro in cui è inserito. Questo è il punto chiave, poi possiamo discutere sulle modalità con le quali la pace si consegue. Noi siamo dell'opinione che non vada solo declamata,

sono ì per difendere la nostra sicurezza, la pace di quel teatro e la sicurezza di quella regione, insieme ai nostri ragazzi presenti in Libano, in Niger, in Gibuti e nelle altre 47 missioni che sono riassunte Se è così - e credo che nessuno dotato di buona fede in quest'Aula possa smentirlo, perché su questo presupposto si fonda la nostra stessa impalcatura istituzionale e costituzionale allora dobbiamo riflettere e ragionare su quali debbano essere le scelte conseguenti. Se guardiamo il perimetro dentro il quale ci stiamo assumendo impegni diretti e precisi,

che la Brigata Wagner ci sarà ancora o no in Africa avrà un impatto diretto sulle rotte migratorie, sul controllo delle terre rare in quel contesto, sulla presenza e sulla pressione della Russia nei confronti di Paesi che probabilmente avrebbero bisogno di una nostra iniziativa politica

siamo presenti all'interno di questa cornice, perché oggi la sicurezza per i nostri cittadini significa stare esattamente su quei punti avanzati. Se è vero, come è vero, che oggi il mercato della logistica è direttamente connesso con la sicurezza delle rotte Est-Ovest, allora si capisce perché i nostri ragazzi stanno in Gibuti: non ci siamo dimenticati

o il fatto che si possa passare in quella zona delicatissima del mondo in una condizione di potabilità, dal punto di vista delle relazioni. Ho fatto solo un esempio, ma ne potrei fare molti altri. Vorrei spendere gli ultimi minuti del tempo che ho a disposizione su un argomento che sarà trattato anche da quest'Assemblea e sul quale vorremmo consigliare particolare prudenza e attenzione, in particolare agli amici e colleghi del Partito Democratico, che ritengono di dover imbastire su questo una posizione ideologica e anche di modifica rispetto al passato: dell'applicazione del *memorandum* tra Italia e Libia. Anche in questo caso non ce la possiamo cavare con battute e slogan generici, non solo perché questi possono soddisfare la platea del momento senza però risolvere il problema, ma anche perché una forza di Governo è tale se dall'opposizione fa

non fa né più né meno che quello che ha fatto il Governo precedente, quindi non si capisce il motivo politico per il quale in quest'Aula si dovrebbe votare contro una proposta di un Governo di segno diverso

esattamente identica alla proposta precedente, in termini politici non si capisce il motivo della differenziazione. Sulla vicenda particolare bisognerebbe anche essere coerenti rispetto all'impalcatura. Il tema della Libia meriterebbe probabilmente una sua articolazione molto più specifica, ma non ne ho il tempo. Intanto l'impianto giuridico della cosiddetta scheda 47 è stato costruito integralmente da Presidenti del Consiglio che facevano riferimento al Partito Democratico e alla coalizione di centrosinistra. Infatti, il Protocollo per la cooperazione tra la Libia e l'Italia è stato sottoscritto a Bengasi il 29 dicembre 2007 (Governo Prodi) e il *memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere interne è stato sottoscritto a Roma il 2 febbraio 2017 (Governo Gentiloni). nella scheda, che è consegnata agli atti, si dicono cose che contrastano anche con le parole che non abbiamo sentito in quest'Aula - forse non ancora - ma certamente in sede pubblica. La relazione governativa sull'attività svolta nel 2022 - attenzione, ripeto, nel 2022 - ci dice che le autorità libiche hanno conseguito, rispetto al passato, una maggiore capacità di efficientamento dei mezzi in dotazione e c'è la necessità di incrementare il grado di preparazione tecnica e la standardizzazione delle procedure manutentive. Per tutti questi motivi, oltre che «per i positivi riverberi in termini di prevenzione e repressione dei traffici illeciti via mare» il Governo Meloni, riprendendo la relazione del Governo Draghi, propone a questo Parlamento di confermare tale misura. Credo che ci sia l'esigenza di una coerenza di fondo, rispetto alla quale chiamarsi fuori esclusivamente per motivi di propaganda politica sia un grave errore politico. Oltretutto - lo voglio dire, in conclusione - stiamo parlando, a fronte di una presenza di militari all'estero estremamente significativa - di una missione che per il 2023 avrà 25 unità di personale - ripeto, 25 unità di personale - della nostra Guardia di finanza, che svolge funzioni di istruzione nei confronti dei militari della Guardia nazionale libica. Lo ha ricordato prima il collega Licheri.

con degli istruttori turchi o russi, avremmo una ricaduta positiva dal punto di vista dei diritti umani, della sicurezza e della libertà? *(Applausi)*. È per questi motivi che serve una coerenza di fondo ed è per questi motivi che voteremo a favore delle missioni internazionali.

approvando sia la proroga di una serie di missioni importanti che prima relatore, senatore Paganella, ci ha ricordato, sia gli ulteriori e nuovi impegni

e anche la vicenda della Libia. Parto dalla vicenda della Libia perché anche in Commissione sono emerse le diverse valutazioni di alcuni Gruppi. Noi, con tutti i dubbi e le perplessità sull'andamento della vicenda libica, riteniamo che sia fondamentale sostenere l'azione della Guardia costiera di quel Paese.

da un lato il richiamo, come dirò tra un attimo, alle ragioni della storia, dall'altro che molte cose hanno una certa apparenza, ma poi la forza della storia sgretola Noi dobbiamo esserci anche nel contesto libico, auspicando che prima o poi quel Paese possa votare e possa avere un Governo, ma tutto è molto lontano. che il vice presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri Tajani annunciava che in Europa - ieri c'è stato l'incontro dei Ministri degli esteri dell'Unione europea

amici miei, la storia è fatta di quello che accade e quindi la Tunisia dovrà completare ancora un suo cammino verso la realizzazione di riforme e del rispetto dei diritti; la Libia si spera che realizzi quello di cui c'è necessità in quel Paese, ma l'Italia o l'Europa non possono rinviare interventi economici in Tunisia o, per quanto ci riguarda - torno così al provvedimento sulle missioni militari - un intervento in Libia anche con la Guardia costiera. Dopodiché, vorremmo uno *standard* di diritti molto più elevato in Libia, conosciamo la complessità ma non possiamo non intervenire per cercare di impedire la moltiplicazione dei viaggi. So che alcuni, forse anche qui in Aula, esprimeranno opinioni diverse, come è accaduto in Commissione,

in quei luoghi, per evitare forme di prigionia inaccettabili, per evitare forme di degrado che ci sono. Sicuramente questo è quello che noi auspichiamo, ma da questo a non intervenire in tali contesti sarebbe contrario agli interessi dell'Italia in un'Europa dove molti si girano dall'altra parte, perché quella nave che poi si è schiantata sulle secche di Cutro non si era mai avvicinata alle coste della Grecia, che pure ha costeggiato e poi abbiamo assistito alla tragedia di qualche tragedia di qualche settimana fa al largo della Grecia, perché alcuni Paesi o si girano dall'altra parte o dicono che sono troppo piccoli, come Malta, per ospitare queste tragedie, ma comunque non fanno quello che l'Italia fa in termini di solidarietà e di accoglienza, che non può però essere illimitata.

di situazioni che moltiplicano la speculazione sulla disperazione, perché sui viaggi della morte molti si arricchiscono e quindi probabilmente nella realtà subsahariana c'è ancora più confusione. altrove ci sono presenze simboliche, ma c'è anche la Wagner, che forse è stata sopravvalutata, ma che manifesta comunque degli interessi verso altre realtà. Le missioni internazionali, in conclusione, sono anche un modo per affermare la presenza italiana. Sono state citate da altri colleghi missioni storiche nel Libano che durano da lungo tempo, la funzione delle nostre Forze armate o dei Carabinieri nella formazione delle forze di Polizia nei Paesi della ex Jugoslavia, le tensioni che ci sono state ancora qualche settimana fa in alcuni Paesi dove etnie, religioni, situazioni diverse si scontrano anche all'indomani di elezioni amministrative. Noi siamo un elemento di ordine e di legalità nel contesto internazionale e dobbiamo vantarcene. È una delle alte funzioni che l'Italia svolge, affermando anche la propria storia,

- intanto porrebbe fine a una discussione un po' troppo politica; dall'altro lato, dimostrerebbe che le Forze armate nelle calamità, nelle emergenze interne e internazionali sono una certezza. Di questo dovremmo ricordarci, quando si fanno le leggi di bilancio, quando si dovrebbe arrivare al 2 per cento del PIL per rispettare gli *standard*

il mio intervento, ci tengo a dire che la storia dimostra che le Forze armate servono non per fare guerre, come purtroppo ha voluto fare Putin, ma anche per portare pace e sicurezza. Nei giorni scorsi la crisi che è scoppiata in Russia ha fatto parlare di cose storiche. Lenin - ha parlato del 1917 e del tradimento del gruppo Wagner, dimostrando che servono Forze armate serie e regolari. Chi fa eserciti di mercenari poi alla fine rischia di trovarseli contro: prima li forma, li va ad arruolare nelle galere, come è successo per la Wagner, e poi quelli tirati fuori dalla galera con un'amnistia per affidargli il lavoro sporco, un giorno o l'altro si ribellano pure al padrone del momento. A questo servono le Forze armate

e che aveva spedito in Ucraina e nel mondo, ha parlato del 1917, quando con la rivoluzione di ottobre, la guerra tra menscevichi e bolscevichi, la pace separata dei russi con i trattati del 1917, si determinò un momento di crisi. Tutto questo, almeno a me, ha fatto pensare che ci sono delle costanti nella storia. Adesso abbiamo una guerra in Europa, con l'aggressione all'Ucraina, che non vogliamo che si estenda. È in corso in queste ore una missione di pace promossa dalla Chiesa: speriamo che abbia successo, anche se pure da Kiev - mi diceva prima il senatore Paroli - i primi commenti non sono dei migliori. Non c'è solo, a volte, l'asprezza, la durezza e il torto di Mosca; a volte c'è anche un po' di comprensibile diffidenza altrui. Noi dobbiamo quindi mantenere uno strumento militare perché non sappiamo che cosa ci riserva la storia. Noi vogliamo la pace, ma l'antico detto recitava: «*si

a evitare che l'Italia sia un approdo di tutte le disperazioni. Ce ne facciamo carico per una quota molto ampia, con grande generosità, ma poi dobbiamo anche pensare alla nostra sicurezza, alla pace e alla democrazia nel mondo. Concludo, signor Presidente, ribadendo che il voto a queste missioni non è un rito periodico, periodico, da fare con distrazione. È un impegno costante, che ci deve richiamare al sostegno allo strumento militare, ringraziando tutte le nostre Forze armate, le donne e gli uomini impegnati in tanti contesti, e ricordandoci che questo pezzo di Stato e di istituzioni va supportato e va motivato in tutti i modi con i contratti, i diritti e tutte le questioni di cui ci occupiamo quotidianamente che fanno parte di un sostegno ampio alle Forze armate, che poi sostengono la libertà, la democrazia, la pace e la sicurezza nel mondo.

mio intervento con un invito ai colleghi e al Parlamento. L'invito è quello di riappropriarsi degli spazi per poter discutere politicamente di ogni singola missione. Nel 2016, con il senatore Gasparri all'opposizione, si approvò la legge quadro sulle missioni internazionali. Secondo me, è già il momento di cambiarla. Abbiamo già dimostrato che non è utile e non si può mai entrare nel merito delle singole missioni internazionali. In questo caso, noi andiamo a votare degli atti di indirizzo per un totale di circa cinquanta missioni internazionali. Credo che non si riesca a cogliere in realtà la reale strategicità della singola missione. Quindi, non si può capire l'impatto che essa ha sulle popolazioni su cui i nostri militari, i nostri uomini, i nostri civili intervengono per stabilizzare le aree.

caso di mettere mano di nuovo alla legge quadro e di riportare nell'alveo del Parlamento la discussione delle singole missioni, nei tempi e nei modi più corretti. Questo era solo per il metodo e per riappropriarci di una nostra prerogativa. Il senatore Enrico Borghi, secondo me, ha svolto un intervento che ha centrato alcuni temi. Noi abbiamo la necessità di intervenire in alcune aree del mondo, non solo per l'instabilità di quelle aree, ma anche, appunto, perché sono parte di una catena di valore o di una catena di approvvigionamento che tutti tacciono, perché l'aspetto economico che sottende talune missioni internazionali è prevalente rispetto all'impatto sulle popolazioni locali e sulla loro incolumità, sull'incolumità di quei popoli. Penso ad esempio a Taiwan. Taiwan è il crocevia strategico di tutta la produzione di semiconduttori del pianeta. Lì esiste un interesse mondiale. Non solo l'Italia, tutto il mondo ha interesse affinché quell'area sia stabile e affinché sia tenuta sicura. Non ne abbiamo parlato. Non abbiamo potuto valutare la possibilità di fare missioni. Noi abbiamo la necessità di garantire tutta la *supply chain* e, aggiungo, anche la *value chain* per quel che riguarda tutte le risorse, dalle terre rare a tutto il resto. Questo dovrebbe essere l'impatto che la nostra scelta politica

mi concentrerò solo sulle quattro nuove missioni perché, come già detto dal senatore Licheri, in realtà sulle altre missioni vigenti da diversi anni noi concordiamo assolutamente.

giustamente ha fatto notare il senatore Enrico Borghi, dicendo che la missione in Libia va abbandonata, quando sappiamo benissimo che abbandonare quella missione produrrebbe probabilmente un'instabilità ancora maggiore e delle ricadute su quelle stesse popolazioni che non ci permetteremo, ovviamente, di far accadere. l'obiettivo politico del Gruppo MoVimento 5 Stelle è che non ci sia nessun militare e nessun civile con incarico militare militare nel territorio ucraino: l'abbiamo chiesto con i nostri ordini del giorno. Abbiamo accennato al fatto che siamo disponibili che i nostri militari, in questo caso sono 80 unità di personale al massimo, possano formare il personale ucraino. Vogliamo che lo facciano in totale sicurezza e che non siano la scusa - per altri, ovviamente - per considerarci belligeranti. In Libia sono tre le unità di personale e, se vado a leggere l'impegno, è più che condivisibile:

ma non la modalità, o quello che perlomeno potrebbe succedere laddove il Consiglio dell'Unione europea decidesse di spostare in terra ucraina i nostri militari e i nostri formatori. Per la Libia «l'obiettivo è di sostenere gli sforzi guidati dalle Nazioni Unite per la pace e di prestare assistenza alle autorità libiche nella creazione di strutture statali di sicurezza, in particolare nei settori della gestione delle frontiere, dell'applicazione della legge e della giustizia penale, al fine di contribuire agli sforzi e a smantellare la rete di criminalità organizzata». Come si fa ad essere contro questo obiettivo? Si può però bisogna considerare le modalità con cui viene attuato, perché se l'obiettivo viene perseguito semplicemente stanziando fondi, potremmo andare a dare fondi permettendo a criminali libici di aprire e chiudere il rubinetto, proprio per ottenere i nostri fondi: questa è la cosa che va evitata. Il tutto sempre nell'ottica di proteggere le popolazioni: in questo caso l'obiettivo principale è proteggere le popolazioni e i migranti, affinché non subiscano quello che l'ultimo rapporto dell'ONU ha mostrato invece essere in atto. Per quanto riguarda il Niger, tutto il territorio africano è di interesse strategico per l'Italia. Niger e Burkina Faso sono in parte confinanti: quell'area è preda di gruppi terroristici. Come si può essere contro una missione che persegue i gruppi terroristici? Non si può, assolutamente. Torniamo però alle modalità: qual è la modalità che il Governo intende perseguire affinché non succeda quello che può accadere in Burkina Faso, in cui al momento ci sono gruppi terroristici che non si offenderanno le autorità del Burkina Faso - definiti da alcuno analisti un narco-Stato, in balia dei narcotrafficanti del Centro America, che lo utilizzano come piattaforma logistica, per gli smerci di migranti, ma anche di droga verso l'Europa? Allora, lì cosa facciamo? Mandiamo formatori e rischiamo di andare a formare militari o comunque personale che potrebbe essere utilizzato da altri esattamente per lo scopo opposto, ovvero per rendere instabile quel territorio? Abbiamo dunque presentato alcuni ordini del giorno, affinché il Governo si impegnasse a perseguire questa linea umanitaria. È evidente che il Governo non può impegnarsi, perché non sa se domani mattina qualche narcotrafficante, con un'ingente o infinita disponibilità economica, andrà a comprare Governi e milizie. È evidente che non può impegnarsi, ma può offrire una rassicurazione, affinché nel momento in cui ci sono le evidenze che ciò sta avvenendo, il Governo torni in Parlamento e riveda le direttive per i nostri militari o riveda totalmente la missione umanitaria.

la protezione umanitaria e gli interessi delle popolazioni e dell'Italia. Io non sono convinto che il Governo abbia le soluzioni in tasca, così come sono convinto che attualmente nessuno abbia soluzioni pronte in tasca. Per questo motivo offriamo un'apertura: il MoVimento 5 Stelle si asterrà sulla prosecuzione delle missioni in essere e si asterrà anche sulle nuove missioni.

quanto tra poco andremo a votare riguarda la proroga delle missioni e delle operazioni già in corso ed ulteriori iniziative di cooperazione e interventi di emergenza già avviati, nonché l'autorizzazione all'avvio di quattro nuove missioni, con l'impiego in media di 7.500 uomini. Annuncio sin d'ora il voto favorevole del Gruppo Lega. L'attuale contesto internazionale è caratterizzato da estrema instabilità, segnato in primo luogo dal conflitto in atto in Ucraina, con ripercussioni di ampia portata sugli equilibri mondiali, sia nell'ambito delle relazioni internazionali che sul quadro economico-finanziario. L'immediata conseguenza dell'invasione russa è stata la volontà da parte di molti Paesi di rafforzare le loro politiche di difesa, a cui aggiungere il rafforzamento della postura di deterrenza e di difesa dell'alleata della NATO, in particolare lungo il fianco Est. Le ripercussioni del conflitto in atto, come dicevo, hanno un'amplificazione del raggio di azione, in quanto si inseriscono in un quadro geostrategico già complesso, in modo particolare nell'area di nostro interesse quale il Mediterraneo allargato, caratterizzato da fattori di instabilità persistenti, da numerose frizioni di faglia sul piano della lingua, del sistema politico-economico, del credo culturale e religioso, delle condizioni climatico-ambientali e dello sfruttamento delle risorse umane. Pensare di guardare alle problematiche della regione mediterranea focalizzandosi solo su di essa, secondo il concetto che più un fenomeno nasce in lontananza da noi e meno sarà influente sulle nostre dinamiche, significa impostare una gestione che ci condanna alla perenne rincorsa degli eventi. Intervenire di volta in volta in maniera reattiva sui sintomi estemporanei, piuttosto che andare ad affrontare la vera causa scatenante la patologia che sovente risiede al di fuori, è frutto di concause. Quello su cui intervengono le missioni internazionali e gli interventi umanitari di cooperazione allo sviluppo va proprio nell'ottica di stabilizzare alcune delle aree più vulnerabili del mondo, in modo particolare le aree di crisi più vicine al nostro Paese, nell'ottica della tutela degli interessi nazionali strategici strategici e vitali della nostra Nazione. Il lavoro svolto dall'Italia per favorire la pace e la sicurezza internazionale è rappresentato dal fatto che siamo il primo fornitore di Caschi blu tra i Paesi occidentali e il settimo contributore al bilancio delle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. Lo facciamo grazie allo sforzo degli uomini e delle donne che servono il nostro Paese, ai quali noi tutti dovremmo dire grazie ogni giorno ed esserne orgogliosi, senza distinguo e senza strumentalizzazione politica da parte di nessuno. Oggi forse, alla luce degli scenari che si stanno avvicendando, dobbiamo fare un salto di qualità, ripensando l'intervento su cui va a lavorare una missione, in modo che possa andare oltre una stabilità ritrovata, ma anche creare le prospettive di sviluppo del Paese dove interveniamo. Proprio in tal senso si è espresso il ministro della difesa, onorevole Crosetto, nel corso dell'audizione sulla delibera missioni 2023 e sulla necessità di affiancare al contributo militare la partecipazione di attori che contribuiscano a realizzare infrastrutture, scuole e università, sistemi agricoli innovativi. Far crescere economicamente, ad esempio, i Paesi del continente africano significa realmente portare a compimento la *mission* che ci ha portato ad intervenire in quei luoghi, non solo a beneficio dell'Italia, ma direi dell'Europa. Significa creare quelle condizioni che permettono ai giovani di pensare a un futuro nel loro continente e non di essere in balia dei trafficanti di esseri umani. Concludendo, Presidente, annunciando il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, vorrei fare un passaggio sul rafforzamento della sicurezza di ambasciate e consolati di fronte alle numerose e gravi minacce subite, con un rifinanziamento del fondo sicurezza del Ministero degli esteri. La sicurezza delle nostre sedi all'estero e del personale che vi presta servizio è garantita dal ruolo encomiabile svolto dai Carabinieri. Proprio su questo, Presidente, vorrei lanciare un appello, che riguarda quanto è avvenuto nel febbraio 2021 in occasione dell'attentato al nostro ambasciatore Luca Attanasio; con lui sono morti il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista. Ebbene, di fatto la procura di Roma ha promosso l'accusa di omicidio colposo e omesse cautele a carico di due funzionari del PAM del PAM (Programma alimentare mondiale); ma noi oggi, come Stato, non ci siamo costituiti parte civile. L'appello che faccio va proprio in questo senso: cercare di rivedere questa posizione e di costituirci parte civile in questo processo, in modo da

Signor Presidente, quando ci si avvicina alle decisioni sugli strumenti principali della politica estera e della politica internazionale del nostro Paese, che danno il senso di come noi investiamo nei principali teatri geopolitici, il Partito Democratico si è sempre assunto le sue responsabilità e lo fa anche questa volta, in continuità con il lavoro fatto dai precedenti Governi. Ricordo il lavoro importante dei nostri Ministri; penso al ministro Pinotti e al ministro Guerini, che per anni hanno guidato quel Dicastero e lo hanno fatto

le donne e gli uomini della Difesa italiana, che tengono alto non solo l'onore del nostro Paese, ma anche quello dell'Europa, delle Nazioni Unite e della NATO, nelle varie missioni internazionali in cui sono impegnati. A loro va la vicinanza, la solidarietà e il ringraziamento del Gruppo Partito Democratico. *(Applausi)*. L'occasione permette di rimarcare, oltre al nostro impegno, anche l'indirizzo politico della nostra politica estera. Parto dall'Alleanza atlantica, dalla NATO, e dal nostro impegno in quelle missioni,

un rafforzamento del nostro impegno in tutto il fianco Est. Questo richiede due ordini in considerazioni. La prima è un sostegno pieno al lavoro che stanno facendo le donne e gli uomini della Difesa italiana, soprattutto in Lettonia, dove siamo presenti da tempo, ma anche con la nostra presenza in

*status* di *battle group* a quello di vera e propria brigata, con un consolidamento della nostra presenza secondo quel tipo di dispositivo. Lo dico perché una riflessione politica dovrebbe vedere la condivisione di tutto il Parlamento; questo è lo stato lo sforzo che abbiamo messo in campo nei passati Governi, sia in quelli a guida PD, sia in quelli nei quali il Ministro della difesa era espresso dal Partito Democratico. Siamo sempre stati molto attenti a compensare il rafforzamento sul fianco Est con un analogo rafforzamento, anzi con una richiesta di definire una vera e propria nuova politica e una nuova strategia per il fianco Sud, per il rafforzamento nel Mediterraneo, che vada oltre la presenza dell'operazione Sea Guardian di controllo e di contrasto al traffico di armi e al contrabbando del petrolio. Ciò anche in termini di sicurezza e di lotta all'infiltrazione del terrorismo di matrice islamica, però in prospettiva a un nostro impegno nel Sahel, quindi a una richiesta di un rafforzamento della NATO anche per quanto riguarda le minacce che arrivano da Sud, dove ormai si è spostata la nuova palestra del fondamentalismo islamico dopo

dopo che abbiamo aperto l'ambasciata, con una missione bilaterale, con l'affiancamento della missione francese Takuba e poi con il ritiro della Francia stessa da alcune missioni che l'avevano vista pagare un prezzo elevato in termini di vite umane.

si è deciso di aprire una missione sul Burkina Faso e vogliamo capire meglio come si andrà a consolidare, se siamo da soli, se siamo insieme all'Unione europea nei vari formati di assistenza e supporto sia ai civili sia ai militari che operano in quei territori in funzione antiterrorismo, per una maggiore sicurezza di quei delle Forze armate. Vogliamo tuttavia anche capire se la NATO è al nostro fianco nel rafforzamento degli strumenti a disposizione, perché adesso gli investimenti sono molto bassi. Abbiamo avuto occasione di parlarne anche con il nostro nuovo ambasciatore alla NATO. secondo punto nelle direttrici della nostra politica estera riguarda la presenza nei Balcani, che è stata ormai consolidata e rafforzata nell'operazione Joint Enterprise. Noi siamo presenti da tempo, dalla fine della guerra civile nei Balcani, abbiamo anche una presenza molto importante in una conformazione europea, in una delle più importanti operazioni nell'ambito dell'Unione europea in Bosnia.

che quei due Paesi trovino un *modus vivendi* anche per evitare incursioni russe in quell'area che, in assenza di una strategia europea chiara, che non può prevedere solo la presenza dei militari ma anche iniziative dal punto di vista politico-diplomatico, rischia di lasciare campo libero alla diplomazia russa in un territorio estremamente fragile e delicato dal punto di vista dei suoi equilibri, anche per le forzature del regime kosovaro in occasione delle elezioni comunali. Su Mediterraneo e Medio Oriente importante il nostro rafforzamento non solo all'interno della coalizione internazionale per la lotta contro Daesh. Essendo *leading nation* della missione NATO in Iraq, Iraq, un nostro rafforzamento a quelle latitudini dimostra che siamo presenti, anche con posizioni di responsabilità importanti, nel tessuto delle missioni e delle operazioni di *peace keaping* e di *peace enforcement* della NATO. Da questo punto di vista dobbiamo alzare le alzare le richieste anche nei confronti dell'alleato americano per avere una maggiore presenza nel Mediterraneo. Lo dico perché noi da soli non ce la facciamo in Libia e nel Sahel, abbiamo bisogno che gli Stati Uniti siano al nostro fianco. Quindi, vanno bene le operazioni che andiamo a rifinanziare e a sostenere. Penso sia importante la nostra presenza negli stretti più delicati (Hormuz e Bab el-Mandeb) e nel Golfo di Guinea, in modo da tutelare gli interessi strategici italiani, soprattutto alla luce del processo di diversificazione energetica. Da ciò deriva l'esigenza di esserci laddove passano i principali flussi di merce e la maggior parte delle forniture di greggio, ma anche del gas liquido che poi viene rigassificato; passano attraverso quei luoghi delicati e strategici dal punto di vista geopolitico e hanno bisogno del rafforzamento della nostra presenza.

della situazione democratica. Anzi, abbiamo assistito a una sorta di *golpe* strisciante: non saprei come altro descrivere quello che è successo in Tunisia, con la sospensione e poi la chiusura del Parlamento, con la sospensione della Corte suprema,

Poi c'è la Libia, su cui ci giochiamo una parte della nostra credibilità. Lo dico da subito: chiederemo la votazione per parti separate per quanto riguarda la proroga delle missioni, mentre voteremo a favore della della risoluzione per le ulteriori missioni. Per quanto riguarda le proroghe, voteremo a favore di tutte le missioni tranne che sulla scheda 47, che prevede il sostegno alla guardia costiera libica con la presenza della nostra Guardia di finanza. È vero quanto diceva il nostro ex collega del Partito Democratico Borghi, ossia che si tratta di una missione che riguarda solo 25 persone, ma io, attraverso il Presidente, voglio ricordare all'ex collega del Partito Democratico Borghi che fu lui a chiederci l'anno scorso astenerci dal votare quella missione e andò addirittura - allora era responsabile della segreteria Letta - dal ministro Lamorgese per chiedere di superarla completamente. Noi non facciamo altro che portare avanti quello che ci chiese il collega Enrico Borghi nella scorsa legislatura: questo a onor di verità. Lo dico perché noi abbiamo una posizione molto chiara. Sappiamo quali sono gli interessi strategici del nostro Paese e sappiamo che dobbiamo garantire la stabilità e la sicurezza di quell'area, che è fondamentale. Ma allo stesso tempo abbiamo l'ambizione di provare a tenere insieme la stabilità e la sicurezza di quel Paese, del Mediterraneo e della Libia, ma anche la tutela dei diritti umani. Infatti, quando ci muoviamo in ambito internazionale, sappiamo che ci portiamo dietro i valori e i principi della Costituzione; e se noi non li rimarchiamo anche nei teatri più complicati e difficili, veniamo meno alla nostra storia, ai nostri valori e ai principi in cui crediamo. È per questo che noi sulla Libia sappiamo per quali missioni votare; sappiamo che siamo a fianco del genio militare che va a fare lo sminamento umanitario, dei nostri medici e infermieri, dei nostri tecnici che fanno *istitution building*, ma vogliamo dare un segnale forte ai membri della guardia costiera libica che hanno violato ripetutamente i diritti umani, si sono resi protagonisti di stupri e violenze. Non possiamo stare zitti e abbiamo il dovere di dire che lì qualcosa deve cambiare.

è un voto tutt'altro che banale quello che esprimeremo tra poco sui due documenti che abbiamo portato all'esame del Senato. Chi mi ha preceduto, in tanti casi ha voluto anche illustrare o specificare alcuni di quei punti che i due documenti contengono. Uno, quello più recente, ci pone di fronte a quattro nuove missioni militari, le altre - sono in 47 in totale - prevedono di fatto il rifinanziamento di missioni in cui l'Italia c'è già. Sono quasi 8.000 i nostri ragazzi - che poi non sono solo ragazzi - in divisa che portano alto l'onore della nostra bandiera, della nostra Patria, ma soprattutto di quell'impegno nobilissimo e umanissimo che sanno assolvere in armi. Ebbene, il voto che daremo questa sera si inserisce in un quadro che è molto diverso da quello in cui spesso si era abituati ad operare. Devo dire che anche il Parlamento, come le istituzioni pubbliche, come la stessa opinione pubblica, era abituato a parlare di missioni di rafforzamento o di mantenimento della pace, bonariamente si parlava di *peacekeeping*,

gli scenari del nuovo quadro geopolitico in cui l'Italia e gli altri Paesi dell'Alleanza si troveranno a operare. Ma sappiamo che il mondo è cambiato davvero.

ma poi c'è un grande scenario di guerra non convenzionale, di guerre ibride che si combattono dappertutto. Devo dire che ho avuto un'esperienza bellissima con la Commissione, anche insieme al senatore Borghi, qualche settimana fa,

Sul fronte Sud di cui parliamo non possiamo non sapere cosa accade. Nel nostro Mediterraneo, affollato purtroppo di profughi, di naufraghi e di tanti morti, sott'acqua c'è un affollamento

la nuova missione in Ucraina in materia di medicina logistica, protezione da agenti chimici, biologici e radioattivi, supporto ingegneristico, cybersicurezza.

che è spinta sul Mediterraneo: da una parte abbiamo l'Africa, con la quale saremo costretti a costruire una grande "politica di cooperazione", perché è fondamentale, perché la massa migratoria si può controllare soltanto così e poi perché ne abbiamo drammaticamente bisogno, perché la crisi russo-ucraina ha aperto la grande questione dell'energia e l'approvvigionamento dell'energia come e dove si fa? C'è il fronte Sud, c'è il fronte Est, c'è il Mediterraneo allargato, ci sono i nostri ragazzi che vengono feriti in Kosovo - ho visto anche loro - che sono lì a difendere i principi di libertà, di giustizia e di rispetto. Con tutta la simpatia che si può avere per il Kosovo, se i nostri militari non fossero lì,

quando ci sono gli snodi della storia, uno non può scherzare, non può fingere di non esserci. Tra l'altro un Paese grande come l'Italia - perché è giusto esserne orgogliosi - quando ci quando ci sono i grandi nodi non può stare fuori, non può fare finta che ciò non avvenga: non ci si può arrangiare a giocare con i gessetti colorati invocando la pace, perché la pace si fa anche, in ogni parte del mondo, mandando i propri soldati, i propri militari, mandando chi ci crede

un Paese serio non può cambiare, non può ondeggiare. Di fronte alle alleanze, di fronte al mondo, di fronte a chi ti sta vicino, di fronte alla tua storia, di fronte al tuo protagonismo, di fronte a quello che sei non puoi ondeggiare, non puoi fare finta di scherzare. Quando, come in questi tempi, che sono drammaticamente difficili, vuoi esserci, devi esserci in ogni teatro e avere anche chi ha il coraggio di farlo. Voglio allora ringraziare questi ragazzi. Tra Tra cinque giorni saranno trent'anni dalla battaglia del *checkpoint* Pasta a Mogadiscio. Fu la prima missione internazionale in cui morirono dei soldati italiani dopo la seconda guerra mondiale.

mi rispose di no, perché era la sua battaglia ed era la battaglia giusta. Le battaglie giuste sono quelle che ogni giorno, in ogni angolo del mondo questi ragazzi, questi uomini e queste donne portano avanti: sono le battaglie per la difesa della libertà, sono le battaglie per la difesa della pace, della giustizia, di chi è oppresso e di chi è aggredito e sono le cose più giuste, più nobili e più belle che alla fine può fare un uomo.

è l'Italia che rappresenta e che sa vivere davvero questa libertà. Guardate le immagini di un nostro soldato che prende un bambino o quelle del nostro soldato che accompagna un bambino che cammina senza le gambe perché è saltato su una mina. Guardate la mano rugosa di un vecchio che si fa accompagnare da uno dei nostri soldati; guardate una donna che a loro sorride. Tutte queste sono le immagini dell'Italia più bella, quella che portiamo in giro per il mondo e che dobbiamo tutti insieme sostenere. Dobbiamo essere orgogliosi di questa Italia, perché porta in alto il nostro onore e la nostra bandiera.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

Signor Presidente, lo abbiamo fatto tante volte e vogliamo farlo anche stasera qui in Aula. Il 27 giugno del 1980, ottantuno persone partirono dall'aeroporto di Bologna su un DC-9 dell'Itavia. Quelle persone non atterrarono mai a Palermo. Nel cielo sopra Ustica, infatti, si svolse una vera e propria azione di guerra nascosta. Aerei di Paesi alleati si levarono in volo per colpire un aereo libico nel quale si pensava fosse il presidente Gheddafi. Ma un missile lanciato da uno di quegli aerei colpì quel DC-9, che precipitò in mare, con quelle persone. Quell'azione di guerra non doveva essere rivelata. L'errore era stato enorme ed enorme era la violazione della nostra sovranità nazionale. Per questo si cominciò a deviare subito, parlando di cedimento strutturale. Era un primo depistaggio. Il resto fu storia di cancellazione di tracciati *radar*, suicidi sospetti di persone che sapevano, di morti altrettanto sospette e di tanti altri depistaggi, come quelli legati alle immancabili piste palestinesi che, come per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto, sono state usate per occultare la verità. Fu un coraggioso giornalista d'inchiesta, Andrea Purgatori, che scavò tra i primi, scoprendo quel muro di gomma abbattuto poi da anni di battaglie e dall'impegno dell'associazione dei familiari delle vittime, di tanti altri protagonisti protagonisti di quegli anni e, soprattutto, dell'indomita Daria Bonfietti, che è stata anche senatrice in quest'Aula. Fu un giudice come Rosario Priore che certificò con sentenza quanto davvero accaduto: altro che cedimento strutturale! Mi avvio a concludere, signor Presidente. Nel corso degli anni, costellati - ripetiamo - da gravi depistaggi, c'è chi non ha mai mollato nella ricerca della verità. Pensate che il presidente Francesco Cossiga, nel 2008, testimoniò e firmò la testimonianza in un tribunale, dicendo testualmente e sotto giuramento che quell'aereo era stato abbattuto da un aereo francese e che volevano colpire Gheddafi, e i servizi segreti italiani avvisarono quel giorno Gheddafi di non volare in quel cielo, a quell'ora, quella sera. Una sentenza definitiva della Cassazione, infine, in sede civile, ha condannato lo Stato italiano a risarcire i familiari delle vittime per non aver saputo proteggere la sicurezza di quel volo, quella sera, in quel cielo sopra Ustica. Infine, signor Presidente,

che allora «oscurò circostanze e responsabilità» e ha aggiunto che «i risultati ottenuti spingono a non desistere, a ricercare» gli ultimi «tasselli mancanti» per il «bisogno di verità e giustizia». siamo stati al museo della strage di Ustica e a abbiamo incontrato Daria Bonfietti. Non cercano vendette, loro e i familiari, ma cercano verità e giustizia, e lo fanno con determinazione. Lo dico a tutti noi: è interesse che ci sia quel timbro, che quel Paese alleato dica: "Sì, eravamo noi: abbiamo sbagliato". È interesse del nostro Paese, della dignità del nostro Paese. Ci hanno provato altri Governi, in passato, senza riuscirci. Non sto dando le colpe, ma chiamiamo il Governo italiano in carica a fare il suo dovere: facciamolo insieme! Chiudere quella ferita, senza vendetta, ma con verità e giustizia, non è un dovere solo verso i familiari, ma è un dovere per l'Italia intera. la scorsa settimana, ancora una volta, i lavoratori Almaviva sono stati costretti a scendere in piazza per veder riconosciuto il loro sacrosanto diritto al lavoro. Ancora una volta mi trovo costretta a denunciare la deprecabile pratica dell'utilizzo della clausola sociale come strumento di ricatto dei lavoratori e, cosa ancor più grave, nell'ambito di commesse pubbliche. Gli "angeli del 1500", gli operatori Almaviva comandati dal Ministero della salute per la gestione del numero verde dedicato all'emergenza Covid, si sono ritrovati a non avere una commessa a cui far ritorno, perché nel frattempo quelle di provenienza erano state cedute, senza che venisse in alcun modo protetto il diritto al futuro occupazionale di oltre 500 persone. Persone e non numeri, che oggi ancora attendono di sapere quale sarà il loro destino, alla fine del 2023. A parte un modesto piano di incentivi all'esodo e alla possibilità di riqualificarsi nel settore dell'IT, che ha riguardato però qualche decina di lavoratori, per la stragrande maggioranza degli operatori non è ancora giunta nessuna risposta dal tavolo di crisi istituito, né relativamente alla riattivazione del servizio 1500, né tantomeno alla conferma che nessuno di questi lavoratori venisse abbandonato al suo destino. La politica nazionale e locale targata centrodestra ad oggi si è riempita la bocca di parole e buoni propositi, senza però portare a casa alcun risultato concreto per questi lavoratori. Adesso, però, si apre un nuovo capitolo con l'avvicendamento di Comdata ad Almaviva nell'appalto Trenitalia, a seguito della dichiarazione, da parte di Comdata, secondo cui ci si troverebbe in presenza del 30-35 per a fronte dei quali sarebbe necessaria una pesante riduzione oraria, con palese elusione della clausola sociale. Dal momento che la società cedente Almaviva applica un ammortizzatore al massimo del 10 per cento, sembra evidente come questo sia un passaggio per eludere nuovamente la clausola, il tutto nel silenzio assordante di Trenitalia, società del gruppo FS, che non manifesta alcun interesse nei confronti dei lavoratori e del servizio di assistenza clienti. Un silenzio surreale, se si pensa che da oltre una settimana vi è uno sciopero totale, con conseguente blocco del servizio, unico strumento dei lavoratori per portare l'attenzione sullo stritolamento della clausola sociale. Basta con questo siparietto. Ribadisco la richiesta al Governo di convocare subito Comdata, Trenitalia e i sindacati per mettere tutti in riga e garantire un integrale rispetto della clausola sociale a tutela del servizio pubblico di assistenza ai clienti della nostra compagnia ferroviaria. Lo Stato, noi tutti, non possiamo restare indifferenti dinanzi a questa ennesima vicenda giocata sulla pelle di donne e uomini, che chiedono solo il rispetto del diritto al lavoro. La legge non può essere calpestata.